L’ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 119, 1004, 1034, 1931 recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

l’individuazione di un territorio contiguo all’area del parco che, nonostante sia esterno al perimetro del parco stesso, venga sottoposto alla governance dell’Ente parco. Non riteniamo cioè opportuno che il regolamento del parco definisca l’esercizio delle attività anche nelle aree ad esso contigue e anche contigue ai siti di importanza comunitaria (SIC) e alle zone di protezione speciale che ricadono anche parzialmente nel perimetro del parco, sottraendo con questo le competenze al Comune e alla Regione.

vigente, il parco, accertati squilibri ecologici, può tentare di ricomporli con prelievi faunistici e abbattimenti selettivi, autorizzando in pratica la caccia. Con la modifica viene invece inserito esplicitamente il divieto assoluto di praticare attività venatorie nei parchi nazionali e regionali ed è pertanto chiara la volontà di proibire anche una eventuale deroga mediante il regolamento del parco.

e del Governo perché anche la 1[a] Commissione permanente, con la nota dell’8 novembre, nel formulare le osservazioni al disegno di legge, afferma che nella procedura di approvazione del regolamento del parco è opportuna la previsione

e non alle Province autonome, di manifestare solo il dissenso non è infatti idonea ad assicurare il pieno esercizio delle prerogative costituzionalmente riconosciute in materia alle Regioni e alle Province autonome. Pertanto, riteniamo che l’emendamento 5.122

perché non condividiamo la disposizione secondo la quale, rispetto alle aree contigue, possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, specialmente se si pensa alla grande estensione del territorio protetto nazionale. Si tratta di un’imposizione di divieti assurdi che non rientrano nella giurisdizione dell’Ente parco. Allo stato attuale - lo sottolineo - la caccia nelle aree contigue viene regolamentata dalle Regioni.

Il paradosso lo voglio sottolineare - è che l’Ente parco non paghi i danni causati dalla selvaggina nelle aree contigue, ma solo quelli causati all’interno dei parchi. senatrice De Petris

5.106 riguarda un argomento che attiene alla vicenda della fauna,

un’unica associazione, in contrasto anche con l’articolo 18 della Costituzione. Quindi, riterrei un elemento di buon senso il nostro emendamento che sopprime tale ipotesi.

il parco consolida i principi della conservazione, compie una serie di operazioni importanti per la tutela del territorio

di chiusura, prevede che a far data dall’approvazione del piano non sono consentiti all’interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso e, a far data dall’approvazione, tali previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti su tutte le previsioni di piani territoriali urbanistici. Al riguardo vi è una vecchia discussione, perché

il numero totale dei capi catturabili o abbattibili, il periodo specifico entro il quale il controllo si attua e i confini precisi e le aree soggette alle operazioni di controllo,

Per quanto riguarda l’emendamento 5.117, esso contiene la richiesta, che viene dal mondo dei movimenti ambientalisti, di una maggiore partecipazione della

il 5.118, con il quale si specifica che tutte le associazioni di enti gestori di aree protette a livello nazionale o regionale saranno rappresentanti istituzionali del settore, proprio attraverso la consulta del parco.

creare discontinuità con la loro funzione. Si chiede, quindi, che le piante organiche dell’Ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle riserve naturali statali finora garantite dal Corpo forestale dello Stato,

Presidente, l’emendamento 5.138 è volto a ripristinare e implementare le capacità e le modalità di gestione economica delle aree protette italiane.

finalizzata alla salvaguardia e alla conservazione delle stesse. Si rendono pertanto imprescindibili misure urgenti e necessarie in grado di garantire agli enti gestori una maggiore autonomia direzionale

parco è chiamata all’elaborazione di un piano economico e sociale pluriennale volto alla promozione di attività che - come meglio specificato nel comma 3 - siano ritenute maggiormente idonee a fronteggiare le condizioni emergenziali in cui versano le aree protette. Tali attività fatto salvo il rispetto della tutela del parco, in attività a carattere ludico o sportivo, nonché in quelle strettamente connesse all’istituzione dei cosiddetti ecomusei. A tale proposito appare opportuno sottolineare come detti ecomusei abbiano negli anni raggiunto notevole maturità e rilievo, rivestendo un ruolo di grande interesse presso il mondo accademico, le le istituzioni locali, regionali e nazionali, le associazioni di categoria, in particolare dell’agricoltura e dell’artigianato, di operatori e soprattutto dei cittadini. Pertanto, questo vasto movimento sociale, culturale e territoriale merita di ottenere un riconoscimento da parte del legislatore e di essere inserito nel programma di valorizzazione delle aree protette tra le altre attività meritevoli di sovvenzioni.

che è attualmente previsto dalla legge n. 394 del 1991. Il provvedimento in esame, infatti, elimina tale silenzioassenso sull’inerzia dell’Ente parco nell’esprimere il parere sugli interventi infrastrutturali, anche per i casi di interventi minori. noi riteniamo che l’inerzia colpevole dell’Ente parco, che attualmente ha sessanta giorni per potersi esprimere, non deve assolutamente determinare la paralisi dei procedimenti amministrativi dell’autorizzazione. Quindi confidiamo nell’accoglimento di questa proposta di emendamento.

Presidente, nel mio intervento di ieri ho cercato di sottolineare come noi fossimo in linea con un’idea di semplificazione, oltre che di miglioramento, dell’utilizzo delle risorse e delle opportunità che le aree protette esprimono.

Vorrei che si riflettesse sul fatto che la semplificazione è indispensabile e che gli stessi Enti parco possono usufruire dei criteri di semplificazione (stessa governance), anche perché molto spesso le strutture di cui dispongono non sono nelle condizioni di esprimere approfondimenti tali da poter, poi, veramente coincidere con le esigenze dei cittadini.

ampliarne la portata, nel senso di rendere giustizia a quella fascia di territorio che si trova a ridosso dei confini del parco e che maggiormente subisce, dal punto di vista dei danni materiali alle attività agricole, l’invasione di razze che sono giustamente protette nell’ambito dell’area dell’Ente parco.

la legge prevede incentivi sia da parte dello Stato, sia da parte delle Regioni; ma ogniqualvolta un cittadino danneggiato si rivolge alla Regione o allo Stato per ottenere questi incentivi si sente rispondere che non esistono fondi nei capitoli di bilancio.

cui chiediamo di sopprimere le royalty per gli impianti a biomasse che vanno contro l’attività agricola.

visto che per il momento si prevede che le royalty siano date soltanto ad attività già esistenti, credo sia necessario crea- re un fondo ministeriale vincolato

di fare una riforma a costo zero. Che cosa si è messo in campo? Si è messo in campo questo meccanismo delle royalty che dovrebbe diventare uno degli elementi per il finanziamento. È vero che la presenza di impianti all’interno delle aree parco deve portare - ed è giusto che sia così - a un risarcimento e a una compensazione ambientale, anche di natura economica, proprio per

Contemporaneamente, però, bisogna fare in modo che questo meccanismo non diventi un elemento di condizionamento dei parchi stessi e degli enti gestori dei consigli

riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all’interno delle aree protette, nonché delle aree contigue,

in quell’occasione facemmo anche una scoperta stupefacente, nel senso che ci accorgemmo che in realtà gli introiti di questa tassa sono bassissimi, ciò che lascia supporre

di entrate da destinare allo scopo, il parere della 5[a] Commissione è stato di nullaosta. Quindi, spostare l’aliquota da un livello ad un altro non cambia nulla.

ho appena ascoltato l’intervento del Presidente della Commissione bilancio, il quale ha detto che non c’è problema se si cambiano le percentuali.

non condividiamo la disposizione che impone delle addizionali a tutti i canoni concessori, alle concessioni idroelettriche, alle attività estrattive, al passaggio di oleodotti e metanodotti, ai beni demaniali, a titolo di contributo alle spese dell’Ente parco per il recupero della naturalità. Peraltro, tale imposizione non riguarda solo le aree interne al parco, anche perché alcune attività sono proprio vietate all’interno dei parchi, ma riguarda anche tutte le aree contigue. Sottolineo che saranno sottoposti alla nuova tassa anche gli agricoltori titolari di impianti a biomasse nelle aree del parco e nelle aree contigue. Si tratta dunque, in ogni caso, di un innalzamento della tassazione che non si ritiene condivisibile, specialmente nel periodo di crisi economica attuale e in considerazione della difficoltà che attraversano le nostre imprese. Confermo quindi il voto contrario

dell’articolo, il 9.103, che cerca di riportare a criteri assolutamente scientifici

problema di dover garantire la tutela della biodiversità e quindi di dover garantire un equilibrio e una gestione molto accurata e oculata della

di interventi di controllo faunistico, anche spinti, questi devono avvenire su iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione e ad opera del personale dipendente, dei

venatoria e il compito di tenere sotto controllo e gestire in modo adeguato la fauna selvatica.

(M5S). Signor Presidente, forse c’è il senatore Russo che vuole chiedere il voto elettronico. Non vorrei anticiparlo. PRESIDENTE. Non lo vedo così convinto.

l’emendamento 26.105, in quanto estraneo all’oggetto del disegno di legge in esame; dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 13.100, 15.0.101 e 15.0.102

nell’Arma dei carabinieri), nonché la proposta 20.101, che reca una delega al Governo senza l’indicazione dei principi e dei criteri direttivi.

questo è uno degli articoli che purtroppo abbiamo intercettato come rispondenti a una logica diversa da quella che intendevamo per

al fine di diminuire il gravame sanzionatorio di alcune situazioni, che non sono certamente penalmente rilevanti, ma sono amministrativamente perseguibili e non certo con questa intensità.

pur considerando che sono passati alcuni anni dall’introduzione della riforma. In un clima in cui, complessivamente,

i pescatori e alcuni operatori economici che vivono ai margini delle aree protette e che, alle volte, possono, anche incolpevolmente, incappare in alcune infrazioni che dovrebbero essere di Per questo motivo abbiamo presentato una serie di emendamenti e, in ordine a questi, attendiamo un chiarimento del Governo per quanto riguarda la gestione di questi episodi da parte delle aree protette.

17.109, potremmo anche prendere in considerazione l’ipotesi di trasformarlo in ordine del giorno.

di struttura giuridica, non solo del provvedimento ma del nostro ordinamento. Da troppo tempo, purtroppo, siamo abituati, come cittadini, a subire conseguenze anche penali derivanti da circolari: per quel poco che ho appreso sui banchi di scuola e di università, nella nostra legislazione una norma penale dovrebbe essere solo norma emanata dal Parlamento e non certo norma decisa da enti

tornassero a essere l’equivalente della trasformazione delle lire in euro, senza aggravi, pur comprendendo il trascorrere del tempo. Come ho detto infatti, ci sono già termini molto elevati di sanzioni, peraltro nei confronti di categorie deboli, come quella dei pescatori, che vivono proprio ai margini della sopravvivenza e dell’equilibrio del bilancio economico delle loro attività.

visto che il senatore D’Alì chiede che_ ci si esprima, ci si esprime: non è previsto l’arresto per l’attraversamento in zona C nelle aree marine protette delle Egadi, ma il rilascio di un’autorizzazione per il passaggio. La condotta penalmente rilevante è quella connessa al rilascio delle reti da strascico durante il passaggio che in ogni caso, per essere segnalata al magistrato, richiede la contestazione in flagranza da parte della capitaneria.

da parte di chi viene eventualmente perseguito, in questo caso anche con l’arresto. Per quanto io sia concettualmente contrario ad applicare

stati recepiti né dal relatore, né dal Governo. In particolare, mi riferisco alla richiesta di istituzione del parco nazionale del Barsento, ovvero in una zona ad alta

potremmo farci sfuggire l’occasione di normare un ecosistema che va assolutamente tutelato e salvaguardato. Pertanto, ritengo che ci siano tutte le condizioni per poter impegnare il Governo affinché tale

salvaguardia attraverso l’istituzione di un’oasi di protezione faunistica. Nel frattempo, le amministrazioni locali di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Putignano hanno provveduto ad individuare ad individuare ed approvare una delimitazione del potenziale parco e la Regione Puglia ha emanato una una normativa consequenziale. Oggi, purtroppo, a distanza di tanti anni, non è ancora operante un regime di tutela. Per questa ragione, propongo sia gli emendamenti, che eventualmente sarei disponibile a ritirare, sia l’ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la necessità di istituire questo parco.

naturale nelle zone del Barsento, assicurando al contempo le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al suo funzionamento». DEGANI, sottosegretario

sull’emendamento 20.101. Il parere è non ostativo, a condizione che nelle disposizione di delega ivi prevista siano inseriti i principi e i criteri direttivi, nel rispetto dell’articolo 76 della Costituzione.

si avvale della possibilità di formulare anche il parere ambientale, togliendo questa prerogativa agli enti preposti, ossia alle sovrintendenze. Durante la discussione generale, abbiamo ascoltato qualche collega dire che le sovrintendenze sono degli impicci alla libera imprenditoria, alle attività che fanno progredire questo Paese.

quando dobbiamo dare l’autorizzazione ambientale perché non ci sono le competenze (e si torna sul concetto di competenze) per concedere quell’autorizzazione ambientale. Avremo, come dire, un manuale di riferimento e ci prenderemo l’ardire di stabilire se le opere previste sono conformi. Io credo che questo sia gravissimo ma, tra l’altro, è in perfetta linea

autorizzazione ambientale semplificata. Vorrei mostrarle la foto di una pavimentazione fatta a Lecce, dove è stato messo asfalto davanti ad una chiesa

si valuta che esse non erano conformi, ma non si può rimediare quando il danno è stato già fatto. Questa non si chiama semplificazione. Stiamo facendo un danno gravissimo al nostro patrimonio culturale

invece stiamo facendo con questo provvedimento che mercifica anche i parchi e le risorse naturali. Lo stiamo facendo con altri provvedimenti. PRESIDENTE.

in accordo con il MIBACT e con l’Osservatorio delle politiche culturali del Ministero, all’interno del quale si

ai parchi di redigere il piano del parco tenendo conto dei piani paesaggistici delle rispettive Regioni. In assenza dei piani paesaggistici (e sono pochissime le Regioni che li hanno), si prendono a riferimento gli articoli del codice Urbani, che determinano i vincoli del paesaggio. Non solo: il parco deve fare la valutazione ambientale strategica, cosa che non era prevista prima.

caso su questo punto, che sta molto a cuore al MIBACT, è stato dato parere favorevole. Volevo tranquillizzare i colleghi sul fatto che non ci sarà nessuno sfregio, nessuna violenza ai beni paesaggistici. Anzi, secondo me, con questo sistema, noi li tuteleremo ancora di più. Sulle competenze, in questi anni, all’interno delle aree protette, sono arrivate le migliori competenze che possiamo avere per quanto riguarda la parte tecnica. tranquilli. Non votiamo nulla di strano. Non c’è la libera uscita ai violentatori del paesaggio. Anzi, c’è maggiore tutela e rigore. Per

Il Senato approva.

Signor Presidente, l’articolo 25 del disegno di legge sulle aree protette reca delega al Governo per l’istituzione del Parco del Delta del Po. L’istituzione di questo Parco non consentirebbe di tutelare adeguatamente le popolazioni residenti in questa splendida area del Paese,

Insieme al collega Amidei ho presentato degli emendamenti per difendere la gente e coloro che da tanti anni, da generazioni, svolgono la propria attività lavorativa all’interno del Parco. b), inserire la seguente: «b-bis) prevedere misure specifiche che tutelino la piccola pesca e la pesca turismo, e un maggior controllo nel tentativo di scongiurare le attività di pesca illegale che contribuiscono alla crisi del settore;». Inoltre, ci chiediamo come verrà regolamentata la caccia nel momento in cui si prevede in capo al costituendo Ente parco, quando le stesse regole sottendono alle norme regionali. regionali. Con l’emendamento 25.101 chiediamo che la sede operativa degli organi del Parco del Delta del Po sia ubicata tenendo conto dell’estensione territoriale e, quindi, nella Provincia di Rovigo. Non si può prescindere dalla peculiarità di un territorio e dalle esigenze dello stesso, nonché dalle attività presenti e future e non si può e non si deve procedere in alcun modo senza prima aver tenuto in debita considerazione la volontà della gente locale che vi abita e opera, direttamente o attraverso le proprie rappresentanze.

dichiarazione di voto.

segue gli incontri che si stanno svolgendo sul territorio con i sindaci e con i rappresentanti di categoria. In primo luogo, vi è la contrarietà assoluta all’ipotesi di parco nazionale. La governance deve rimanere in capo ai territori. Non è accettabile il concetto che il costituendo parco unico sia prodromico alla nascita di un parco nazionale, come ha affermato il collega Caleo nella sua relazione al provvedimento. Ricordo che la trattativa avviata con la Regione Veneto e il Governo partiva dal concetto di legge speciale sul Delta e presupponeva un’ipotesi di coordinamento gestionale tra i due parchi e non un parco nazionale. Vi è contrarietà netta all’ampliamento della superficie del parco e all’introduzione di nuovi vincoli sul territorio. Il parco deve essere interpretato non come camicia di forza, ma come elemento di sviluppo e promozione del territorio e delle attività umane in esso esistenti, in particolare la pesca, la vallicoltura, l’agricoltura e la caccia. Deve essere dunque chiaro il ruolo necessario delle attività umane per la vivibilità, la manutenzione e la produttività del Delta. Essendo la parte veneta del parco quella di maggior valore naturalistico e avendo peculiarità del punto di vista ambientale economico e sociale del tutto del tutto distinte da quella emiliana, dovrà necessariamente avere adeguata rappresentanza e propria autonomia gestionale in seno al costituendo ente. Vogliamo poi capire se e quante risorse saranno destinate dal Governo al predetto parco; dovrà, infine, esserci il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali e delle categorie produttive. Non verrebbe mai accettato un parco che risulta il frutto della sola visione delle associazioni ambientaliste e che scavalchi i rappresentanti istituzionali ed economici del territorio. dunque che la decisione finale della Regione Veneto sul decreto legislativo del Governo sarà presa alla luce dei precedenti aspetti e dopo aver sentito il territorio. Per il Gruppo Lega Nord-Autonomie deve rimanere un punto fermo che nessuna decisione dovrà essere imposta dall’alto e senza il pieno coinvolgimento della popolazione. La Regione si farà garante di questo. Alla luce di questi nostri rilievi, nonché preoccupazioni, il Gruppo Lega Nord-Autonomie esprimerà un voto di astensione sul’articolo 25 in attesa dell’esercizio della delega da parte del Governo per l’espressione di un parere finale complessivo.

esprimendo il voto convintamente favorevole sui contenuti dell’articolo 25, che è frutto innanzitutto di ritardi

culturali, hanno convenuto sulla necessità, ma soprattutto sull’opportunità di rilanciare questo strumento e questa occasione di sviluppo sostenibile dei territori. Nell’articolo 25 non si fa altro che ribadire questo aspetto: pertanto,

vale a dire la delega potrà essere esercitata con l’intesa delle due Regioni. Dunque le preoccupazioni che il collega Arrigoni illustrava mi sembrano quantomeno infondate rispetto al contenuto vero dell’articolo.

III. Discussione del documento: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009